Restano confermati gli argomenti previsti dal calendario della settimana corrente. Alla luce dell'*iter* dei lavori presso le Commissioni riunite 5ª e 6ª, la discussione del decreto-legge concernente misure di carattere fiscale ed economico, già prevista per la seduta odierna, potrà avere inizio giovedì 26 o, direttamente, lunedì 30 settembre, alle ore 16. Resta confermato che giovedì 26 settembre, alle ore 10, avrà luogo la votazione per l'elezione di due componenti del consiglio di amministrazione della RAI. Il calendario della settimana potrà essere integrato con un'informativa del Governo sulla detenzione in Italia di Maysoon Majidi. All'inizio della seduta odierna un rappresentante per ciascun Gruppo interverrà sulla situazione in Medio Oriente. L'Assemblea tornerà a riunirsi, come anticipato, lunedì 30 settembre, alle ore 16, con l'eventuale seguito della discussione del decreto-legge in materia di misure di carattere fiscale ed economico. La prossima settimana verrà altresì discusso, dalla sede redigente, il disegno di legge in materia di insegnamento della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'educazione civica. Saranno discussi, inoltre, i disegni di legge in materia di manifestazioni di rievocazione storica e norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e, ove concluso dalle Commissioni, il disegno di legge in materia di morte medicalmente assistita. Nella settimana dall'8 al 10 ottobre, con sedute a partire dalle ore 14 di martedì, saranno discussi il Piano strutturale nazionale di bilancio di medio termine e il disegno di legge in materia di durata delle operazioni di intercettazione. alle ore 9,30, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e del 18 ottobre 2024. Nella settimana dal 15 al 17 ottobre, inoltre, saranno discussi i disegni di legge in materia di introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio e in materia di contrasto alla surrogazione di maternità. Giovedì 26 settembre, nonché il 3, il 10 e il 17 ottobre si svolgeranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

per l'*escalation* in atto al confine fra Israele e Libano, dove la conflittualità latente e a bassa intensità dei mesi scorsi sta sfociando in una vera e propria guerra.

Ormai la situazione sembra fuori controllo. Stiamo parlando, del Libano, dove la risoluzione 1701/2006 delle Nazioni Unite è stata violata da entrambe le le parti, dove ci sono decine di migliaia di sfollati da entrambe e le parti e dove soprattutto sta aumentando il numero di morti. Negli ultimi due giorni, gli attacchi delle forze di difesa israeliane hanno prodotto già più di 600 morti, dei quali 50 bambini: una carneficina che deve essere fermata in ogni in ogni modo. Oltre alla preoccupazione, nell'area, per l'*escalation* e per l'impatto geopolitico, in un equilibrio già fragile, messo a dura prova da uno scontro devastante a Gaza, dove la tragedia umanitaria continua e dove, appunto, le diplomazie internazionali non riescono a trovare una via per la liberazione degli ostaggi e la cessazione

un'informativa in tempi rapidissimi al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa; al Ministro degli affari esteri per capire quali azioni il Governo sta mettendo in campo insieme ai *partner* europei, i *partner* atlantici e le diplomazie con cui abbiamo rapporti in Medio Oriente per

La preoccupazione è enorme: gli Stati Uniti hanno appena diramato una nota in cui chiedono a tutti i loro cittadini di abbandonare velocemente il Libano. Sono stati sospesi i voli della stragrande maggioranza delle compagnie aeree. Insomma il clima è davvero drammatico e ci aspettiamo che in tempi rapidissimi il Governo possa essere qui in Aula per informarci, spiegare qual è la situazione, che tipo di iniziative diplomatiche intende intraprendere e soprattutto rassicurarci, per quanto possibile, sulla situazione dei nostri militari nell'area.

ritenuti concordi nel chiedere la presenza in Aula dei due Ministri degli affari esteri e della difesa, proprio per riferire a tutta l'Assemblea sulla situazione

riteniamo importantissimo che il Ministro degli affari esteri ci dica se la postura è cambiata, se ha colloqui con Israele e se intende fare pressioni su di esso affinché muti

una nuova postura nel sacrificare le vite umane tramite la nuova tecnologia cercapersone. A noi sembra terribile quello che sta accadendo e ovviamente speriamo che vada a placarsi.

tutti i giorni aumenta i bombardamenti e la guerra in quell'area, con un'*escalation* che rischia di andare fuori controllo. Rischiamo davvero la guerra mondiale,

il Governo Netanyahu, perché ha una responsabilità fortissima nell'*escalation* su questo terreno. È quindi opportuno intervenire con forza e dire esplicitamente basta:

accolto questa istanza), di poter dedicare l'inizio dei lavori dell'Assemblea di questa settimana al tema delle drammatiche notizie che ci stanno giungendo in questo momento dal Medio Oriente, significativamente dal confine fra Libano e Israele. Riteniamo sia non solo giusto e doveroso, ma indispensabile che tutti i Gruppi parlamentari si pronuncino e che il Governo venga impegnato nel riferire immediatamente, nelle forme e nelle modalità che la Presidenza riterrà di dover organizzare nel più breve tempo possibile. che il ministro Tajani è impegnato in queste ore all'Assemblea generale dell'ONU e che il ministro Crosetto è in missione istituzionale, quindi non pretendiamo di imporre una calendarizzazione immediata. Poniamo però il tema dell'esigenza di una strutturazione dei nostri lavori, in Commissione o in forma congiunta con le Commissioni affari esteri e difesa della Camera, per consentire che il Parlamento approfondisca e che il Governo riferisca su un tema così delicato e così complesso, non solo per le questioni di merito, rispetto alle quali sappiamo che la polveriera attorno alla vicenda libanese si stava accendendo da tempo. Abbiamo ancora in mente le drammatiche immagini dei bambini drusi uccisi nel bombardamento che ha colpito un villaggio in Galilea; abbiamo in mente le centinaia di migliaia di cittadini israeliani che sono stati costretti ad abbandonare tutta la fascia nord del loro Paese, a seguito del pervicace e costante bombardamento messo in atto da Hezbollah. Noi rischiamo di rincorrere le agende quotidiane dell'informazione, ma nel mentre si realizzava il dramma di Gaza si andava anche configurando una costante attività di bombardamento del nord di Israele da parte di Hezbollah. Quindi siamo giunti alle drammatiche immagini di queste ore che impongono

dedico a questo gli ultimi due minuti che mi sono concessi - non dobbiamo dimenticarci che in quel teatro abbiamo una responsabilità come Paese. Paese. Esattamente in quel contesto sono presenti 1.256 nostri militari all'interno della missione UNIFIL, che dal 1978, sotto l'egida delle Nazioni Unite, assicura una forza di interposizione. Proprio nel mese di agosto i militari della Brigata Sassari hanno sostituito gli alpini della Taurinense; inoltre sono presenti i nostri Carabinieri e la nostra Aviazione dell'Esercito con sei mezzi. Insomma, abbiamo una responsabilità che non è solo politica, ma è anche operativa. Quindi, abbiamo bisogno di sapere dal Ministro della difesa come stanno i termini della questione, come si intende intervenire per tutelare e mettere in sicurezza i nostri militari nella circostanza e, più in generale, per assicurare un'iniziativa politica, diplomatica ed istituzionale per andare nella direzione del contenimento di una situazione che è esplosiva. Utilizzo gli ultimi trenta secondi per dire che già ieri in Libano avevamo 2 milioni di sfollati provenienti dalla Siria, su una popolazione che non supera i 7 milioni. Oggi abbiamo un milione di libanesi che si sta spostando dalla zona Sud verso Beirut: non ci vuole molto a capire quale può essere la conseguenza di tutta questa vicenda. Il quadro giuridico è molto preciso: è la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1701 e dobbiamo mettere in campo tutte le azioni per la sua concretizzazione.

noi ovviamente ci associamo alla richiesta della presenza del Governo, in particolare - certamente del Ministro della difesa - del ministro degli affari esteri Tajani, che - voglio sottolinearlo - sicuramente parteciperà, compatibilmente con il calendario vigente, a questa ulteriore iniziativa di confronto con il Parlamento. Il ministro Tajani ha infatti sempre adempiuto, forse statisticamente molto più di altri suoi predecessori, al confronto sia con le Commissioni, sia con le La situazione in atto è certamente meritevole della massima attenzione per tutto quello che, ancora una volta, si sta determinando nell'area del Medio Oriente, nel Libano, a Gaza. Tra qualche giorno - lo voglio dire fin d'ora - ricorrerà - ricorrerà l'anniversario di un evento che ha determinato questa situazione. Nessuno dimentica che quello del 7 ottobre è stato un tentativo di sterminio di un popolo: non è stato un episodio di guerra, ma è stato l'attacco a case, a famiglie, a donne, ad anziani, a bambini nei loro domicili, a giovani che

entrati in questa drammatica fase perché, altrimenti, faremmo una valutazione sbilanciata. Tra pochi giorni, credo il 7 o 8 ottobre, anche qui in Parlamento, ci saranno iniziative per ricordare a un anno da quei drammatici e tragici quello che è successo, ossia un tentativo di sterminio, che poi innesca­ - ahimè - quello che è accaduto. Il ministro degli affari esteri Tajani in queste ore è all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Se leggete le cronache, ha presieduto poche ore fa ci sono fusi orari diversi, ovviamente - la riunione dei Ministri degli esteri del G7, che si è occupata anche di altri aspetti, perché c'è la crisi del Medio Oriente, c'è il problema dell'Ucraina, degli approvvigionamenti per l'Ucraina con l'inverno che si avvicina. E poche sere fa il ministro degli affari esteri Tajani si è recato a Parigi per una riunione dei cinque Ministri degli esteri principali.

una rilettura, una reinterpretazione della Bibbia e osservavamo, commentando quel libro che tutti poi leggeremo, come ahimè, fin dai tempi della Bibbia, le stesse zone, gli stessi popoli, gli stessi conflitti, gli stessi drammi si rinnovano da millenni. Questo non vuol dire che ci si debba rassegnare a questa tragedia, che è antica, affonda le sue radici nella storia e che deve essere affrontata ponendo fine alla morte dei palestinesi e anche, però, al delirio di chi parla di un unico Stato dal fiume al mare, l'espressione che sostanzialmente prevede che dalla Giordania alle sponde del Mediterraneo Israele non dovrebbe più esistere. Ed è ancora il linguaggio con il quale alcuni volevano celebrare il 5 ottobre a Roma, con una manifestazione di senso contrario, l'anniversario del 7 ottobre, come se fosse una vicenda da celebrare. È quindi giusto intervenire e dialogare, cosa che il Ministro degli affari esteri fa, nei limiti di quello che le ragioni della storia ci fanno capire. Ma è giusto che ci sia anche un confronto nel Parlamento, come c'è sempre stato. Anche le ultime le ultime iniziative vedono il Governo italiano protagonista, con la Presidente del Consiglio, ovviamente, all'assemblea annuale dell'ONU. Quindi l'Italia è ben presente e attiva e credo che anche la nostra Presidenza del G7 sia stata retta sin qui con grande capacità

per il modo in cui rappresentano l'Italia nel mondo e tutelano le ragioni della pace tra i popoli, sia che si tratti dell'Ucraina, sia che si tratti del Medio Oriente e di tutti gli altri scenari dei quali ci dimentichiamo, talvolta, perché dal Sudan ad altri posti ci sono guerre dimenticate che creano dolori, lutti e massacri ai quali forse dovremmo dedicare più attenzione.

Commissione affari esteri e difesa del Senato, hanno richiesto un'informativa dei ministri Tajani e Crosetto per avere informazioni su quello che sta avvenendo in Libano. La preoccupazione di tutti - e anche noi della Lega ci uniamo in questo

io ho avuto modo di vedere personalmente e che già stava soffrendo di una crisi economica devastante. Oggi a tale crisi economica devastante si va a sommare quella che è in pratica una nuova guerra. È una polveriera, quella del Medio Oriente, che - come

a inizio settembre hanno effettuato una donazione di beni di prima necessità alla popolazione. Quindi, un contingente italiano in una missione di pace è da tempo presente, e oggi più che mai mai noi italiani dobbiamo ribadire il concetto di essere portatori di pace in un momento delicato come quello attuale. *(Applausi)*.

vorranno venire in Aula, non ci sarà alcun problema da parte nostra. Confermo quello che ha detto il senatore Gasparri rispetto a un'interlocuzione con i ministri Tajani e Crosetto che, in questo periodo assai particolare e sicuramente non particolarmente felice per la situazione internazionale, hanno comunque sempre dato al Parlamento una priorità di comunicazione molto intensa. Dopodiché non credo che sia questa la sede per affrontare l'argomento, proprio perché abbiamo capito che prossimamente ci sarà una possibilità di confronto proprio con il Governo e con i Dicasteri più indicati. Su questo mi limito a sottolineare, rispetto a quello che ho sentito, che invece è abbastanza palese, scritto e determinato che l'Italia non partecipa al finanziamento

ma per operazioni premilitari. Questa è una decisione presa. La sensibilità italiana sul punto è sempre stata chiara: se, da un lato, è vero che la tragedia del 7 ottobre, gli attacchi terroristici messi in atto dai terroristi di Hamas il 7 ottobre hanno determinato anche in parte quella reazione che oggi prosegue, è altresì vero che il presidente del Consiglio italiano, onorevole Giorgia Meloni, è stata l'unico *leader* occidentale, alla fine dello scorso ottobre, a essere presente a Il Cairo al primo *summit* di pace; e ciò proprio per dare una testimonianza diretta rispetto a un protagonismo dell'Italia nel Mediterraneo, che appunto fa sì che la nostra Nazione abbia delle peculiarità, dei particolari interessi e una particolare sensibilità per tutto ciò che avviene in Medio Oriente. È stata riportata da alcuni colleghi che mi hanno preceduto la la specificità del nostro rapporto con il Libano; una missione, quella italiana, che dal 1979, senza soluzione di continuità è presente nella terra dei cedri ed è presente nella missione UNIFIL a Sud del Libano, sulla cosiddetta Blue Line, quel confine amministrativo, ma non formalmente politico, che divide il Sud del Libano con il Nord di Israele; ma è presente anche con una missione esclusivamente italiana a As-Samayah ed è presente con una forza di addestramento per le polizie locali a Beirut. Quindi, è chiaro che l'Italia ha tutta una serie di sensibilità e interessi particolari su questo. Sono convinto e non ho alcun motivo per dubitare che

poter riferire alla Presidenza che c'è una larga condivisione sulla necessità di un aggiornamento in Parlamento da parte dei Ministri competenti sulla situazione in Medio Oriente. Sarà ovviamente cura di questa Presidenza riferire in modo tale che si possa pensare a un inserimento di tale punto nel cospicuo e denso calendario che abbiamo concordato poc'anzi. Corre l'obbligo di un'integrazione su quanto esposto prima, relativamente alla votazione per l'elezione di due componenti del consiglio di amministrazione della RAI, prevista per giovedì 26 settembre, alle ore 10: dopo la chiama, le urne rimarranno aperte fino alle ore 13.

altri morti. A causa del cosiddetto temporale autorigenerante, che scarica una quantità di acqua che fino ad ora nessuno ricordava in quella zona - siamo in provincia di Pisa, al confine con la provincia di Livorno, dove poche ore prima, nel tardo pomeriggio i Comuni di Castagneto Carducci e San Vincenzo erano stati colpiti dal medesimo fenomeno il Comune di Montecatini Val di Cecina ha purtroppo subito gli effetti di quella massa di acqua che si è riversata all'interno del fiume Sterza. Purtroppo, oltre ai danni materiali che sono molto ingenti, questa mattina già dalle prime ore ero in contatto con il prefetto di Pisa e i sindaci dei Comuni interessati, tra cui il sindaco Auriemma del Comune di Montecatini Val di Cecina - sono purtroppo decedute

Vigili del fuoco e volontari per trovarli. Tutto il nostro pensiero va alla famiglia straniera che era in vacanza presso il Comune di Montecatini Val di Cecina, al padre e alla madre che hanno perso il loro piccolo. Il pensiero ovviamente va a tutte le vittime dei numerosi

Ci stringiamo attorno alla comunità che in queste ore vive una nuova disgrazia sul proprio territorio. Ci auguriamo che non riaccada, anche se le cronache